Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 giugno. A partire della seduta pomeridiana di oggi, proseguirà l'esame del disegno di legge sulla istituzione del Sistema nazionale delle Agenzie ambientali e saranno discussi i disegni di legge in materia sanitaria e sull'assistenza dei disabili gravi. Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, provvedimenti sull'introduzione del reato di depistaggio, sul contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, mozioni sulle concessioni demaniali marittime e contro la corruzione negli appalti. Nella seduta pomeridiana di giovedì 26 maggio si svolgerà il *question time* con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'Aula non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno, in vista del primo turno delle elezioni amministrative. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da martedì 7 giugno con l'esame del decreto-legge recante misure a favore degli investitori di banche in liquidazione, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione delle ratifiche delle Convenzioni del Consiglio d'Europa per il contrasto al terrorismo

di quanto già chiesto negli scorsi giorni in quest'Aula, ovvero dell'introduzione del DASPO per i corrotti, dell'introduzione della figura dell'agente provocatore, dell'agente sotto copertura,

terza questione.

dell'informativa sull'agguato nei confronti del Presidente dell'ente Parco dei Nebrodi. E, quindi, non possiamo votare qualcosa che è già in calendario. Inoltre, anche la discussione

fare un'analisi del disegno di legge che ci accingiamo a votare. Il provvedimento che stiamo discutendo in questa sede istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, e comprende norme che disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente stesso. A tale Sistema viene attribuito il compito di monitorare lo stato dell'ambiente e della sua evoluzione, tenendo sotto controllo i fattori di inquinamento e fornendo materiale informativo ai diversi livelli istituzionali sempre in tema di salvaguardia dell'ambiente.

Le Agenzie hanno iniziato a confrontarsi fra loro e a misurarsi omogeneamente, spesso attraverso un ruolo di coordinamento centrale svolto dall'agenzia nazionale ISPRA,

quindi, dobbiamo essere in grado di dare risposte chiare, trasparenti e tecnicamente ineccepibili. Il provvedimento, tuttavia, non riuscirà a dare queste risposte perché presenta alcune lacune. Mi riferisco - ad esempio - alle questioni legate all'ARPA. Il disegno di legge oggi in discussione descrive nel dettaglio le attività e le funzioni assegnate all'ISPRA, ma non è altrettanto esaustivo nel chiarire le funzioni dell'ARPA. Si trasferisce all'ISPRA la facoltà di determinare i livelli essenziali e indispensabili delle prestazioni tecniche e ambientali, le cosiddette LEPTA. Queste ultime costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale e rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie, al fine di assicurare una adeguata e uniforme attività del Sistema nazionale. Tuttavia, visto che la scelta dei LEPTA è condizione necessaria sulla quale verrà basato l'intero Sistema nazionale, e quindi anche tutte le attività collegate all'ARPA, si rende necessario che a tale determinazione partecipino pure le Agenzie regionali. Sono questi alcuni dei limiti che l'attuale disegno di legge presenta e che mi auguro in futuro si possano correggere. Per avere un sistema organico ed efficace della rete delle Agenzie su tutto il territorio nazionale, sarebbe necessario - e questa è un'altra criticità riscontrata - individuare le modalità di reperimento di risorse, ma il senso di tale provvedimento decade completamente nell'attuale disegno di legge, non si prevede l'utilizzo delle risorse necessarie per mettere in atto la riorganizzazione del Sistema delle agenzie ambientali. anche dopo il parere della Commissione bilancio del Senato, ha introdotto la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, vanificando, di fatto, tutto il lavoro svolto e svuotando di ogni significato l'intero provvedimento. Una corretta riorganizzazione avrebbe avuto bisogno di risorse, che avrebbero permesso di disporre di una struttura in grado di integrare le competenze dei vari enti e di far confluire in essa le capacità per dare risposte al Paese. Su questo punto la maggioranza non ha fatto abbastanza e bisognerebbe fare di più. Manca il coraggio di alcune scelte importanti e soprattutto il coordinamento con alcune norme che quotidianamente incidono sulla vita dei cittadini e sulle imprese. Il provvedimento non risolve il problema centrale del coordinamento tra le Agenzie e tutti gli altri enti che oggi sono istituzionalmente impiegati nella ricerca e nella protezione ambientale. Il nuovo Sistema non potrà portare a una maggiore integrazione delle informazioni e soprattutto dei dati, al fine di prevenire la deturpazione dell'ambiente. Non vengono definite le condizioni grazie alle quali l'Agenzia nazionale potrà essere parte attiva negli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. A mero titolo informativo si segnala che nel 2016 l'Italia comincerà a pagare salate sanzioni all'Europa per i gravi ritardi nel rispetto della direttiva comunitaria che prevede, da oltre dieci anni, la messa a norma dei sistemi fognari e depurativi. Questo non lo diciamo noi, ma lo afferma Mauro Grassi, responsabile della struttura di Palazzo Chigi #italiasicura, che si occupa di sviluppo delle infrastrutture idriche e di dissesto idrogeologico, affermando, lo stesso, che il 15 dicembre scorso la Commissione europea ha comunicato al Governo che, nei prossimi mesi, proporrà alla Corte di giustizia europea l'importo delle sanzioni. La situazione italiana delle acque reflue, nel frattempo, è da terzo mondo. Il problema riguarda sistemi fognari e depurativi di 1.025 agglomerati, ossia di 2.500 Comuni. Peraltro, il provvedimento non chiarisce nemmeno l'aspetto legato al coordinamento tra l'Agenzia nazionale e le guardie ambientali, che in molte Regioni hanno assunto le funzioni della vecchia polizia municipale, e la sezione dei carabinieri. Soprattutto non si dice dove verranno fatti confluire i militari

rimane sempre un passo indietro, sprecando una grande occasione. In ogni caso, apprezziamo molto l'impegno di molti di noi nel cercare di approvare una riforma migliore possibile e per questo, come Conservatori e Riformisti, ci asterremo.

come già detto in discussione generale, il disegno di legge che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito da una struttura centrale e 21 Agenzie organizzate in 200 sedi operative sul territorio, presenta aspetti condivisibili perché mira a stabilizzare alcune questioni lasciate in sospeso con la legge n. 61 del 1994. Il Gruppo Lega Nord condivide l'obiettivo di assicurare un'omogenea disciplina per le attività delle ARPA, che invece, fino ad oggi, sono state esercitate in maniera differente nelle diverse aree del Paese. La situazione è ormai ventennale e vede alcune Agenzie, soprattutto quelle al Nord, svolgere controlli serrati e applicare norme rigide alle imprese e altre addirittura sorvolare su evidenti situazioni illegittime

è anche il divieto per le attività di consulenza delle Agenzie in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete, per evitare palesi situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale. Un altro aspetto di garanzia rappresenta il principio di rotazione del personale delle ARPA incaricato degli interventi ispettivi nei singoli siti o negli impianti, ciò al fine di assicurare la terzietà dell'intervento ispettivo e l'imparzialità di giudizio. Positiva è la previsione di realizzare un sistema a rete dei laboratori accreditati. Condivisibile è, infine, la realizzazione e la gestione del SINA, sistema informativo nazionale ambientale, che si avvale di poli territoriali, avremo l'ARPA, detentore ufficiale del dato ambientale, facendo così cessare l'assurdo che ha portato il Parlamento, per anni e sino ad oggi, a legiferare sulla base dei dati di Legambiente. Ma ai sopraelencati aspetti positivi si affiancano diverse criticità. Innanzi tutto non è immediata l'operatività di molte norme contenute nel provvedimento, operatività che è invece subordinata all'emanazione di futuri

dell'invarianza finanziaria, restano congelati sulla carta, con ciò pregiudicando l'efficiente ed efficace erogazione dei servizi. Nonostante l'ISPRA poi non abbia un'adeguata struttura organizzativa che, in questi anni, ha palesemente mostrato profonde carenze operative, le viene assegnato un ruolo rafforzato in termini gerarchici, assumendo anche funzioni di coordinamento della programmazione delle Agenzie regionali attraverso la somministrazione di un programma triennale. Non ci piace assolutamente che ISPRA predisponga da sola questo programma triennale delle attività del Sistema nazionale senza il contributo e la partecipazione delle Agenzie che sono chiamate solo alla fine a esprimere un parere. Inoltre, sempre per ISPRA, il mancato intervento sui compiti di "ricerca", che vengono lasciati permanere con un accavallamento delle competenze con i nuovi compiti di coordinamento delle Agenzie regionali, certamente aggraverà gli attuali problemi sulla struttura organizzativa in termini di razionalizzazione è relativa al meccanismo dei LEPTA che, ancorché utile, per come è definito limita fortemente l'autonomia operativa e organizzativa delle Agenzie regionali. Se i LEPTA sono definiti in modo indipendente dalle differenti pressioni presenti sul territorio e, invece, sono rispondenti unicamente alla standardizzazione di azione e costi, si rischia di ledere gravemente le esigenze specifiche dei territori, perdendo cognizione di specifici fenomeni. L'Italia è lunga e diversa e presenta diverse pressioni ambientali. Infine, sulla scelta del personale ispettivo riteniamo sia profondamente sbagliata la previsione di un regolamento basato solo sul principio del merito, che introduce criteri criteri soggetti e discrezionali. Dovevano essere anche considerati, non solo in un ordine del giorno ma in un emendamento, i criteri di professionalità, competenza, conoscenza e formazione. Quelle sopra evidenziate sono solo alcune delle criticità che mi hanno portato ad avanzare proposte emendative, prima in Commissione e poi qui in Aula, purtroppo bocciate. bocciate. In conclusione, condividevamo fosse necessaria ma questa riforma della disciplina del Sistema nazionale a rete delle Agenzie ambientali verrà ricordata per essere un provvedimento centralista, che si allontana dal principio federalista: un provvedimento pasticciato, monco e, dunque, inefficace. È centralista per il negativo ruolo dato all'ISPRA, Istituto che da troppo tempo - ricordiamocelo - con le profonde carenze operative ha dimostrato di poter un provvedimento pasticciato perché, per l'arroganza della Ragioneria generale dello Stato, è stato riempito di clausole di invarianza finanziaria, dopo gli articoli e ora anche nella parte finale del testo; un'incomprensibile imposizione dei tecnici di Via Venti Settembre, cui non ha fatto fronte una necessaria ed auspicata determinazione della politica, soprattutto quella rappresentata dal nutrito drappello di senatori del Partito Democratico nella Commissione bilancio di Palazzo Madama,

dettavano condizioni profondamente diverse. E poi rimarrà un provvedimento monco, con tante criticità, delle quali ho sottolineato solo una parte per brevità di tempo. Insomma, sono stati persi due anni da quell'aprile 2014, La relatrice Manassero, che comunque ringrazio, unitamente al sottosegretario Degani e ai colleghi della Commissione ambiente e territorio, ha detto che con il provvedimento è stato fatto un passo in avanti. A nostro avviso, è stato fatto un passettino ed è mancata la volontà di introdurre un miglioramento efficace. Senza le risorse umane e soprattutto economiche per fare monitoraggi e controlli, non si va lontano. Resterà dunque difficile prevenire e contrastare le ecomafie, ma soprattutto i nuovi reati ambientali recentemente introdotti con la legge n. 68. E intanto - lo ricordo - il Corpo forestale dello Stato è stato smantellato; intanto le cronache e le inchieste fanno emergere sempre più l'esistenza di inquinamenti e disastri ambientali creati in passato, cui altri se ne aggiungeranno, visto che sempre più aziende, per la profonda crisi economica con il fenomeno della delocalizzazione (che il *premier* Renzi non contrasta), chiudono l'attività, lasciando sul terreno problemi e fideiussioni, presentate e difficilmente escutibili, tali da non consentire il perseguimento del principio «chi inquina paga». È per questi motivi che, pur apprezzando lo spirito della riforma, il Gruppo Lega Nord e Autonomie si esprimerà con un voto di astensione sul provvedimento. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo di Miglianico, in provincia di Chieti, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. Benvenuti, ragazzi.

onorevoli colleghi, le Agenzie ambientali delle Regioni e delle Province autonome in Italia sono in tutto ventuno e sono state istituite attraverso leggi regionali, in un lasso di tempo cha va dal 1995 al 2006.

è caratterizzato però da una forte disomogeneità ed anche da arretratezza normativa. Infatti, le Agenzie regionali, pur presenti in tutte le Regioni, versano in uno stato di generale difficoltà, dovendo operare con risorse inadeguate e scontando problemi di coordinamento fra di loro e anche con l'ISPRA. Inoltre, queste svolgono compiti differenti a seconda delle diverse aree del Paese e possiedono capacità di intervento non sempre sufficienti e strutture spesso inadeguate. Dal punto di vista tecnologico, poi, non tutte le agenzie sono in grado di svolgere le medesime attività e paradossalmente i loro laboratori sono finanche troppi e non ci sono risorse umane ed economiche a sufficienza per mantenere i livelli di qualità e di efficacia. A fronte di questa disomogeneità, le Agenzie regionali hanno necessità di fare sistema. In primo luogo, hanno necessità di confrontarsi sulla gestione di problematiche che spesso sono sovraregionali

risparmi; insomma, di realizzare sinergie per migliorare sensibilmente la qualità del lavoro tecnico-scientifico. Quindi, si capisce come questo raccordo sia fondamentale e come sia assai importante che le Agenzie regionali possano assumere atti tecnici sulla base di protocolli dì lavoro omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, anche per garantire ai cittadini la necessaria parità di trattamento nelle diverse Regioni. Di fatto, quindi, il provvedimento che oggi esaminiamo non fa altro che istituire formalmente quel sistema che già le Agenzie regionali da tempo pongono in essere, seppur nella forma di un coordinamento spontaneo. Certamente si tratta di un provvedimento sentito come necessario e rappresenta sicuramente una buona opportunità per far sì che il sistema di protezione ambientale faccia veramente il tanto atteso salto di qualità. In particolare, con questo disegno di legge vengono definite chiaramente le funzioni e le competenze delle Agenzie, che saranno svolte in maniera omogenea in tutte le Regioni. D'altronde le funzioni di conoscenza dello stato dell'ambiente, come pure quella del controllo delle pressioni ambientali, unitamente alla costante attività di ricerca, necessaria per essere aggiornati su temi e problematiche, specie quelli riguardanti gli impatti ambientali sulla salute, su cui è maggiormente focalizzata l'attenzione dei cittadini, sono i punti-chiave della *mission* delle Agenzie regionali, cui vanno aggiunte le attività di divulgazione della conoscenza e di educazione ambientale, fondamentali per il mutamento degli stili di vita delle nuove generazioni. Uno degli aspetti più qualificanti della riforma, costituito dalla qualificazione dei dati ambientali e dalla previsione dei cosiddetti LEPTA, cioè i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, è sicuramente positivo. Essi costituiranno il riferimento obbligatorio perché i piani di attività delle singole Agenzie ambientali contemplino un livello minimo omogeneo

dovranno essere definiti attraverso un Catalogo nazionale dei servizi, anche al fine di armonizzare le risorse finanziarie. Questo aspetto non è indifferente, dal momento che oggi sempre più il benessere della persona passa da un collegamento stretto tra ambiente e sanità, poiché non vi è dubbio che le condizioni di salubrità delle matrici ambientali producono effetti certi sulla salute umana. Dal provvedimento oggi in esame scaturisce anche un altro dato positivo che è quello del rafforzamento della rete informativa nazionale, gestita da ISPRA in collegamento con le Agenzie regionali. Si tratta di un rafforzamento importante per la collaborazione che l'ISPRA darà alla pubblica amministrazione a tutti i livelli, per la raccolta, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati. Il provvedimento interviene però anche su un altro punto importante, quello dell'organizzazione dei laboratori di analisi ambientale. Con la creazione di una rete nazionale dei laboratori sarà infatti più facile armonizzare su scala nazionale i servizi che questi rendono, nonché realizzare forti economie di scala, oltre all'innalzamento e all'omogeneizzazione del livello tecnico-scientifico e delle attività di controllo, di conoscenza, di analisi e di valutazione. Allo stesso modo è lodevole lo sforzo di dare una migliore sistemazione al settore dei controlli ispettivi. Quello dei controlli sull'ambiente è sempre stato un tema assai critico. Da più parti ci siamo lagnati che le norme a monte non bastano, se poi il sistema non riesce a garantire controlli efficaci sul rispetto delle norme a protezione dell'ambiente. Proprio in queste carenze di controlli molto spesso l'illegalità e il malaffare cercano spazi di impunità. Pertanto, anche sul fronte degli ufficiali di polizia giudiziaria, il provvedimento prevede una proposta equilibrata, che introduce nell'ordinamento una norma precisa in capo all'ISPRA e alle Agenzie, per cui tra il personale possono essere individuati quei dipendenti che opereranno con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il meccanismo di nomina *ad hoc* esclude qualunque automatismo nella declinazione della norma: questo per noi è un fatto positivo. Ancora, all'articolo 15 del provvedimento riscontriamo con favore la previsione di un principio comunitario tante volte richiamato anche in questa Aula, che è quello del «chi inquina paga». Si prevede, infatti, che le spese riguardanti il rilascio di pareri sulle autorizzazioni ambientali e lo svolgimento dei successivi controlli siano sempre posti a carico dei gestori degli impianti e delle attività interessate. Questa previsione permetterà di non far gravare sui cittadini i costi delle verifiche di impatto ambientale soprattutto sugli impianti industriali, che sono - come tutti sanno - potenzialmente più inquinanti e da cui deriva una maggiore esigenza di effettuazione dei controlli. Certo non ci sfugge, cari colleghi, che una riforma così importante per le sfide ambientali del futuro, necessita di uno sforzo di coordinamento e di armonizzazione con tutta la normativa ambientale che è stata prodotta più di recente. Mi riferisco al collegato ambientale, alla disciplina

Sul punto nutro qualche perplessità, dal momento che un organismo che nasce come ente di ricerca, di fissazione di protocolli tecnico-scientifici e di controllo ambientale non so fino a che punto

senza che siano previste le risorse necessarie, dal momento che - come ho ricordato all'inizio - ci risulta che a tutt'oggi le Agenzie ambientali operino in carenza di risorse finanziarie adeguate. Mi auguro pertanto che il percorso non venga impoverito o reso inattuabile strada facendo, perché questo costituirebbe senza dubbio una

Signor Presidente, sottosegretario Degani, colleghi, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e in tale ambito la nuova disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono scelte che devono essere valutate in termini di sistema, perché è in tale contesto che il controllo pubblico ai fini della tutela ambientale assume i requisiti necessari ad adeguate politiche di sostenibilità ambientale. Qualità e salvaguardia dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, sviluppo sostenibile, tutela della salute quale ragione attiva nel contrasto ai fattori di inquinamento sono gli obiettivi strutturali che devono essere perseguiti e che richiedono un organico sistema di *governance*: sistema di governo nel quale ricerca, elaborazione e conoscenza dei dati scientifici siano condizione di sostegno e di coordinamento delle funzioni e delle competenze ai diversi livelli istituzionali e amministrativi interessati. Si persegue in tal modo un ulteriore sviluppo dell'integrazione degli interventi sia che si consideri le politiche di prevenzione attraverso un maggior monitoraggio dei fattori di rischio sia che si operi per adottare e confrontare accordi di programma e misure congiunte di intervento per la tutela ambientale. Riconoscimento e valorizzazione delle competenze degli organi territoriali, con particolare attenzione per noi al ruolo delle autonomie speciali, accordi quadro tra i Ministeri della salute e dell'ambiente dall'altra parte, sono la base per la definizione di scelte operative nazionali e regionali che devono riguardare servizi e prestazioni ai fini della protezione civile, sanitaria e ambientale.

e di determinare i livelli essenziali di prestazione in materia di ambiente (i LEPTA, cui già si è accennato). La definizione della personalità giuridica e dell'autonomia dell'ISPRA, seppure sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, in termini di organizzazione, ricerca e gestione; la semplificazione degli enti componenti attraverso la loro fusione nel nuovo ed unico istituto; l'individuazione di standard minimi e omogenei in ordine di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale della salute, concorrono alla formazione di modelli sinergici ed efficaci. Imparzialità delle attività di controllo e prevenzione e piena diffusione dei dati e delle conoscenze sono opportunamente considerati come condizioni vincolanti, che si integrano fra loro, della logica di rete cui è ispirata l'istituzione dell'ISPRA a livello nazionale, e la valorizzazione del ruolo delle Agenzie ambientali regionali e provinciali sul territorio alle quali sono riconosciuti pari livelli di autonomia scientifica ed amministrativa. È auspicabile che l'adozione del decreto ministeriale relativo alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, tramite la definizione di un Catalogo nazionale dei servizi, avvenga, avvenga, come indicato dal provvedimento in esame, entro un anno dall'approvazione di questa legge. Ciò è fondamentale in ordine al previsto programma triennale che sarà riferimento essenziale per l'attività delle diverse Agenzie ambientali territoriali. L'integrazione dei diversi livelli di conoscenza e delle funzioni nazionali e territoriali, che il provvedimento pone quale obiettivo indispensabile e uniforme per le Agenzia ambientali nell'ambito dell'ISPRA, presuppone che occorra ispirarsi a criteri e parametri al tempo stesso strutturali e flessibili, che consentano un'effettiva valutazione e comparazione dei dati e dei risultati raggiunti sul territorio. È una visione dinamica del sistema di *governance* ambientale che rappresenta la garanzia concreta per un equilibrato e non pregiudiziale confronto in merito a ciò che potrebbe e dovrebbe essere uno sviluppo economico-sociale sostenibile. Per tali ragioni, l'istituzione dell'ISPRA, l'integrazione e la semplificazione delle diverse Agenzie ambientali regionali e provinciali costituiscono una risposta efficace di sistema alla logica opposta, che abbiamo conosciuto, della proliferazione degli enti e dei livelli di controllo. Anche sotto questo profilo si opera in una prospettiva europea di relazione in modo che nei nostri Paesi vi sia più armonizzazione anziché pianificazione, flessibilità anziché rigidità, diffusione delle conoscenze piuttosto che gerarchie e obiettivi astratti, autonomia delle Agenzie ambientali sul territorio entro però un sistema nazionale che esalti sinergie e coordinamento, e si doti di effettivi modelli di valutazione

pari ruolo partecipazione e responsabilità, perché è questa la condizione necessaria a considerare la dimensione globale dell'ecosistema da tutelare. ed è un modello di riferimento sul piano nazionale ed europeo, come autonomie speciali abbiamo operato per la tutela dell'ecosistema alpino e con tali requisiti la salvaguardia ambientale è fattore di sviluppo e di crescita.

Eppure, questo è un provvedimento che riteniamo sostanzialmente positivo, perché credo non fosse più rinviabile la riforma di tutto il settore delle Agenzie ambientali, sia nazionali che regionali, che non fosse più rinviabile una riforma che portasse all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente cui affidare le funzioni di indirizzo, di coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio e ricerca, disciplinando anche l'ISPRA come uno degli istituti fondamentali in questo sistema.

che i controlli ambientali e il monitoraggio dovessero rimanere affidati alle strutture che facevano capo alle ASL, ai presidi multizonali, e chi riteneva fondamentale invece creare un sistema con le agenzie. Questo Questo sistema ha dato vita in questi anni ad una serie di criticità che si sono manifestate soprattutto per la profonda disomogeneità tra funzioni, risorse e meccanismi delle varie Agenzie regionali, con molte differenze tra Nord e Sud a tra le varie Regioni. Questo è stato uno degli elementi più critici in un Paese che - vorrei ricordarlo - scopre con ritmo impressionante la compromissione di aree vaste del proprio territorio, disastri ambientali e inquinamenti molto diffusi (penso agli ultimi dati allarmanti sui pesticidi). Alla domanda se fosse necessaria una riforma strutturale abbiamo ritenuto di dover dare una risposta positiva.

come livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale e perché viene stabilito che questi livelli debbano essere attuati dal sistema nazionale nel suo insieme, ISPRA e Agenzie regionali.

alla richiesta da parte dei cittadini di essere informati, di avere informazioni serie e non discutibili. Il diritto all'accesso riguarda la salute; l'impatto ambientale e i livelli di inquinamento e monitoraggio hanno un effetto diretto sulla vita delle persone e sul diritto alla salute. Questi aspetti sono strettamente connessi. Devo dire, per la verità, che su questo piano, sul garantire un accesso e livelli di informazione più capillari, forse avremmo potuto fare uno sforzo maggiore. E qui arriva il secondo punto.

oggi noi andiamo a votare, per l'appunto, una riforma che, a causa della richiesta della clausola d'invarianza finanziaria, non vede messo in campo alcun tipo di risorse. È vero che all'articolo 15 è previsto il principio chi inquina paga, per cui

con delle risorse sia per il personale sia per il funzionamento. La questione della creazione del Sistema nazionale, che è un passo in avanti, non può rimanere una riforma che alla fine rischia di non essere attuata o che avrà delle difficoltà proprio per la mancanza

che si è sempre occupato e si è specializzato nella repressione e nella prevenzione dei reati ambientali. Non vorremmo che oggi anche questo importante passo in avanti che facciamo sulla riforma

della tutela ambientale, della salvaguardia del nostro patrimonio e della tutela della salute dei cittadini non può più essere considerata una questione secondaria su cui non si stanziano le risorse e su cui non si fanno investimenti per quanto riguarda il personale stesso. è uno degli elementi fondamentali se veramente vogliamo fare in modo che il nostro Paese possa riprendere un percorso e un cammino di sviluppo e di benessere. la riforma della Agenzie ambientali si protrae da otto anni. Noi sosteniamo da tempo una semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza per le imprese. La riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, e l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente sono le tre condizioni necessarie non solo per contrastare l'illegalità ambientale, ma per tutelare le imprese più innovative e per garantire al nostro Paese uno sviluppo di qualità. Inoltre, la crescente preoccupazione dei cittadini riguardo al tema ambiente e salute richiede una risposta da parte delle istituzioni al passo con i tempi. Conoscenza, trasparenza, professionalità sono caratteristiche fondamentali per cui la gente possa riconoscere negli organi tecnici quella autorevolezza indispensabile per avere fiducia e per sentirsi tutelata nel bene supremo che è la propria salute. La costruzione di fatto di un sistema delle Agenzie di protezione ambientale diventa, quindi, una priorità assoluta. La loro costituzione, con la legge n. 61 del 1994, ha segnato un traguardo importante, ma ora diventa indispensabile andare oltre. Non partiamo da zero. Già oggi le Agenzie e l'ISPRA contano oltre 200 sedi al servizio del Paese, 600.000 campioni analizzati ogni anno, quasi 100.000 operazioni tra ispezioni e sopralluoghi, oltre 73.000 istruttorie e pareri, più di 11.000 operatori coinvolti. Sono numeri importanti. Aumentano le attività e diminuiscono i costi per il cittadino. Nel 2012 le Agenzie regionali hanno ricevuto 563 milioni di euro di finanziamento pubblico da parte di Regioni e Province, l'80 per cento circa dai Fondi sanitari regionali. Numeri - dicevo - importanti, ma che non garantiscono un'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei controlli necessari. Le Agenzie del Sud sono sicuramente quelle più in difficoltà, nonostante spesso le emergenze ambientali riguardino proprio quelle Regioni: l'ILVA di Taranto, la terra dei fuochi, l'Isochimica, Bellolampo, Malagrotta, Bussi. Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del sistema dei controlli. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme, di assoluta importanza; si intende anche quella complessa attività di monitoraggio e raccolta dati che serve per migliorare il grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali. Si tratta di avere a disposizione dati certi, scientificamente validati, prodotti da organismi tecnici autonomi, che consentano di decidere al meglio per il bene delle nostre comunità. Non c'è territorio oggi nel Paese dove, rispetto alla costruzione di un qualsiasi tipo di impianto, non vi sia conflittualità sociale; una conflittualità spesso dovuta alla scarsa fiducia dei cittadini verso le istituzioni politiche e amministrative, ma anche verso quelle tecniche, purtroppo, sempre più accusate di essere asservite alle decisioni della politica. Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA; definiamo in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, chiediamo più professionalità a chi dovrà dirigere queste organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità competenti, assolutamente indipendenti e scientificamente validi. Si costruisce un vero e proprio sistema a rete coordinato dall'ISPRA. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, che oggi sono lasciate alla buona volontà delle persone. Si mettono in rete i numerosi laboratori provinciali, si integrano le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determinano determinano livelli di prestazione tecnica ambientale uniformi per tutto il territorio nazionale, per cui vengono definiti livelli di tutela ambientale di base, uguali in tutto il Paese. Definire procedure autorizzative uguali per la stessa tipologia di impianti

possono proliferare e altri in cui questo non è permesso. Avremo finalmente un sistema i cui dati saranno considerati ufficiali. Troppo spesso si citano per convenienze, a volte strumentali, numeri che provengono dagli organismi o professionisti più vari. Le Agenzie regionali trovano in questo schema più autonomia e integrano le conoscenze. Già oggi in queste organizzazioni abbiamo eccellenze di grande livello scientifico. Un'attenzione particolare merita il tema ambiente e salute. Il rispetto dei limiti ambientali e un efficiente sistema di controlli sono, di fatto, attività di prevenzione sanitaria. Questa è la ragione per cui sempre più stretta dovrà essere la collaborazione tra il Sistema e l'Istituto superiore di sanità, un altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno, che finalmente consideri l'ambiente non solo il principale bene comune da tutelare, ma anche una grande opportunità per ritornare a crescere.

l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente modifica l'attuale sistema delle agenzie ambientali, ridefinendo il rapporto tra le ARPA e l'ISPRA. L'ISPRA assume un ruolo più chiaro di coordinamento tecnico e di programmazione delle attività del sistema agenziale che si intende sviluppare in modo uniforme a livello nazionale.

vediamo come le Agenzie sono disomogenee. Come è stato già detto da qualche collega, al Nord vi sono dei buoni sistemi di controllo, mentre al Sud delle Agenzie assolutamente sgangherate; vi potrei parlare della Basilicata, della Campania, della Puglia, della Sicilia,

il Governo? Ha imposto in Commissione un emendamento di invarianza finanziaria, dettato

Il testo avrebbe tutte le potenzialità per rendere maggiormente trasparente, credibile e forte il sistema dei controlli ambientali e l'attuazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali su tutto il territorio, rafforzando i sistemi di partecipazione, l'interazione delle banche dati con l'inserimento di capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nonché con attività di supporto all'individuazione e qualificazione del danno ambientale.

il giusto contrappeso alla pur necessaria e tanto acclamata semplificazione, che però da sola, senza controllo, significa caos e arbitrio. È la legge del più forte a danno dell'ambiente e della giusta impresa. Come si realizza tutto ciò, vale a dire un Sistema un Sistema nazionale efficiente e autonomo, senza finanziamenti adeguati? Non parliamo di soldi a pioggia a cui siamo contrari anche noi, essendo assolutamente per la razionalizzazione della spesa pubblica, non per aumentarla, quindi non parliamo di soldi che devono finire nelle

che pesa fortemente sul territorio, grazie ai suoi 180 milioni di *royalty* annui e ai contratti con l'indotto per lo smaltimento dei reflui che solo con la società Tecnoparco ammontano a 5 milioni l'anno. Di contro abbiamo trovato un'ARPAB che strapagherà pure i suoi dirigenti con 150.000 di euro l'anno, ma che non ha mezzi, strumenti e uomini capaci di fronteggiare i controlli, che non ha neanche la possibilità di informatizzare i propri faldoni, di catalogarli, di un topolino spaventato e sgangherato, funzionale al gigante ENI. Eppure il problema dei finanziamenti alle agenzie è vecchio, presente da quando è nato

La nostra proposta del Fondo unico ambientale, che pure è stata accettata con un ordine del giorno, avrebbe dovuto essere introdotta nel provvedimento in discussione, perché poteva essere la giusta chiave di svolta per finanziare tante opere di tipo ambientale che il nostro Paese aspetta da tempo. se è vero che il sistema nazionale delle agenzie relative ai pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e i successivi controlli saranno a carico dei e che le spese relative alle attività connesse all'autorità giudiziaria saranno a carico del Ministero della giustizia, le ARPA hanno la necessità di un'autonomia forte, quindi di un finanziamento che ne garantisca l'indipendenza di gestione per tutti i numerosi ambiti di sua competenza. Noi sappiamo che, per quanto riguarda le voci di spesa, tutto dipende da cosa politicamente si vuole finanziare. Questo Governo ha già dimostrato tante volte che l'ultimo pensiero è l'ambiente; l'ha già dimostrato con il ministro Madia, che ha disperso il Corpo forestale dello Stato. Sappiamo come si è comportato con l'ILVA: dopo dieci decreti-legge

la vita e la salute dei cittadini di Taranto per gli effetti nocivi dell'ILVA. Noi voteremo sì a questo provvedimento, che ci appartiene, ma ci porteremo a casa un bel frigorifero di classe A++ senza avere la possibilità di attaccare la spina, in attesa che - a breve il Movimento 5 Stelle vada al Governo e si facciano i necessari collegamenti elettrici. il provvedimento di cui si tratta è stato approvato alla Camera due anni fa, nell'aprile 2014. Ora si riprende questo testo senza la minima possibilità di apportare modifiche, ancorché necessarie. Infatti, durante l'*iter* in Commissione ambiente del Senato la sola modifica ammessa è stata l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria. In merito a questa scelta non condivisibile ho presentato un emendamento soppressivo - ovviamente respinto - sostenuto dalla seguente motivazione: come è possibile concepire una riorganizzazione e una razionalizzazione delle agenzie, senza destinare le risorse necessarie a tale scopo? Adottare un provvedimento di tale portata mantenendo la neutralità finanziaria significa rendere nullo e inefficace l'obiettivo che si intende perseguire, quantomeno nella fase iniziale, quella più delicata, del primo avvio del nuovo assetto, per il quale occorre prevedere e provvedere ai mezzi finanziari utili all'istituzione del Sistema nazionale. È necessario sottolineare che neppure durante l'*iter* in Commissione è stato possibile, per volontà della maggioranza, migliorare l'impostazione alla base del provvedimento, la quale, di fatto, crea una struttura centralista, che non tiene conto delle diverse *performance* ambientali riscontrabili a livello territoriale, in particolare regionale. Consideriamo elemento di elevata criticità del provvedimento la sua struttura dirigista, che vede l'ISPRA al di sopra di tutto. L'ISPRA, secondo la nuova impostazione, viene posto come un soggetto sovraordinato che fruirà - lasciatemelo dire - del dogma dell'infallibilità ambientale. Sono numerose le disposizioni del disegno di legge in cui si riscontra questa criticità, a partire dal secondo comma dell'articolo 1, per andare, poi, all'articolo 3, lettera *c)*, ultimo periodo, in cui viene stabilito che gli elementi conoscitivi individuati dall'ISPRA costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito riteniamo che questa norma sia poco ragionata e ragionevole, in quanto non si prevede quali possano essere le conseguenze di una eventuale, motivata e necessaria deroga da parte delle pubbliche amministrazioni. Infine, va citato l'articolo 13, comma 2, in cui si dichiara che il Consiglio del Sistema nazionale - il quale, si noti, è presieduto dal presidente dell'ISPRA - esprime il proprio parere vincolante, tra le altre cose, sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. Cosa si intende e come si definisce la natura tecnica di un provvedimento? È un termine talmente vago, indeterminato ed impreciso che può includere qualsiasi cosa che abbia anche la minima attinenza con la protezione ambientale. Non è conveniente, a nostro avviso, che in una legge ci sia una locuzione così ambigua che prefigura l'emissione di un parere vincolante; a tal fine occorre intervenire su questo punto, affinché si abbia una definizione univoca che non lasci margini così ampi di incertezza. Un ulteriore elemento di criticità appare la disposizione in materia di modalità di finanziamento, contenuta nell'articolo 15, la quale prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, sono a carico dei soggetti gestori - tra questi i privati - le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli, anche con riferimento alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinanti. Tuttavia, la disposizione nulla dice, e riteniamo sia un ulteriore punto molto critico, sui criteri da adottare per quanto riguarda le tariffe future, salvo rimandare a quelle già applicate dalle agenzie a livello regionale o provinciale, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali che verranno in seguito stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. Da un lato, dunque, le modalità di finanziamento che rimangono in via di definizione, per cui tuttora incerte, dall'altro l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria. Sembra quasi che fino ad oggi sia stata generata spesa improduttiva che non ha portato ad alcun risultato. È come girare su se stessi per tornare al punto di partenza. Quindi, delle due l'una: o la maggioranza ha introdotto la clausola di invarianza consapevole, senza dichiararlo, che i margini di efficientamento nel funzionamento di ISPRA sono rilevanti e tali da permettere il recupero di risorse in quantità necessaria a supportare il nuovo sistema, oppure vi è la volontà di non far decollare il nuovo modello. Nell'uno e nell'altro caso, meglio sarebbe stato se la maggioranza avesse fornito indicazioni chiare in merito senza ripetere il solito *refrain* "dichiaro ma non faccio, vorrei ma non si può fare", che caratterizza pertanto molti punti dell'azione di governo. Oltretutto, ulteriore criticità, è piuttosto inverosimile che il sistema nazionale a rete riesca a dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, quali il livello qualitativo e quantitativo di attività che dovrà essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale. In questo modo non si tiene conto delle differenti esigenze territoriali e delle *performance* raggiunte a livello regionale. Il fine di istituire un sistema a rete è condivisibile anche se non è opportuno, a nostro avviso, accentrare tutte le attività in materia di protezione ambientale all'ISPRA, che già è un ente iperburocratizzato che conta più dipendenti, 1.250 circa, del Ministero dell'ambiente e che un domani rischia di ingessare ogni iniziativa "alternativa" in materia ambientale. Se oggi l'ISPRA rappresenta l'elemento di coesione del sistema (così si legge nel sito dell'ente), pur nel rispetto delle realtà territoriali, domani il rischio è quello di eliminare uno degli elementi più importanti del sistema che governa la protezione ambientale, ovvero l'attenzione e la valorizzazione delle realtà territoriali, come dimostrato da numerosi studiosi del settore e da autorevoli prese di posizione basate sulla realtà dei fatti. Un ulteriore punto critico del provvedimento in questione attiene al personale ispettivo. In particolare, la disposizione secondo cui il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato non pochi dubbi. Lo si legge anche nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, in cui si sottolinea che la disposizione presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive, In conclusione, Presidente, condividiamo l'obiettivo alla base del disegno di legge, ovvero quello di istituire un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con il riordino, unito però ad un'azione di valorizzazione delle ARPA. Non siamo convinti dell'approccio, seguito dalla maggioranza, di negare sostanzialmente ogni modifica migliorativa alla quale avevamo inteso fornire il nostro fattivo apporto; errore che, a nostro avviso, comporta l'approvazione di un testo tuttora caratterizzato da criticità che, se non superate, rappresenteranno rappresenteranno un intoppo serio alla concreta ed equilibrata realizzazione della rete delle Agenzie. La nuova legge porta con sé nodi non sciolti, che vanno dall'entità delle risorse alla*governance* del nuovo sistema, alla trasparenza richiesta nei rapporti con i gestori privati di sistemi e di impianti. Su tutto ciò, in conclusione, si staglia l'approccio ipercentralista caro al Governo Renzi, che perde l'occasione di valorizzare pienamente quanto esiste ed è efficiente nella logica dell'omogeneizzazione verso il basso, senza riuscire a rafforzare il sistema delle Agenzie e senza riuscire ad esprimere l'auspicabile coordinamento sinergico. Per queste ragioni ed altre, che i colleghi De Siano e Scilipoti hanno ben evidenziato in sede di discussione generale e in occasione dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

esprimendo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la solidarietà politica, oltre che la vicinanza umana (dopo che lo hanno già fatto i colleghi Lumia e Caleo questa mattina), al commissario del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, colpito nella notte da un attacco mafioso, che solo grazie

di scoperchiare il sistema dell'affitto dei pascoli a famiglie mafiose, che ricevevano i contributi europei per colture biologiche mai realizzate. Ciò che è accaduto è un segnale di allarme forte, un grido che dimostra come i parchi siano un presidio di legalità fondamentale. Oltre ad essere strumenti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del territorio, essi sono un baluardo e un ostacolo agli interessi delle ecomafie. Chi lavora e se ne occupa in prima linea, al di là del ruolo, svolge un compito difficile, spesso non considerato, che lo Stato dovrebbe valorizzare e proteggere maggiormente. Onorevoli colleghi, la riforma di cui stiamo discutendo oggi in quest'Assemblea è in discussione nel Paese da ben otto anni e, come Partito Democratico, ci siamo fatti carico di portare a termine questo lavoro, dando una risposta organica, in grado di sottrarre alla discrezionalità e all'incertezza, oltre che alle differenze territoriali, le imprese e i cittadini. Il lavoro fatto alla Camera, con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge, e poi qui al Senato poteva indubbiamente essere più breve. Aspettare così tanto tempo per un parere sull'articolo 81 della Costituzione e chiedere soltanto l'invarianza di spesa delle norme, peraltro già garantita in più un articoli, ci ha lasciati un po' interdetti, non solo perché ciò costringe il provvedimento a tornare in terza lettura alla Camera per una modifica inerziale, ma perché, per essere condivisa, avrebbe dovuto essere intesa ed interpretata prima, sul complesso del provvedimento come uscito dall'altro ramo del Parlamento, ed eventualmente - come diceva anche la collega De Petris - migliorata in alcune sue parti anche qui. Ci auguriamo tuttavia che i colleghi della Camera contengano al minimo i tempi di esame del disegno di legge e lo facciano diventare legge dello Stato al più presto. Voglio ringraziare la relatrice, la collega Patrizia Manassero, per la conduzione del lavoro, assieme ai colleghi del Gruppo PD in Commissione ambiente e a tutti i colleghi della Commissione, a partire dal presidente Marinello, per la tenacia e la pazienza mostrate nel raggiungimento di questo obiettivo, assieme ovviamente al sottosegretario Degani e al ministro Galletti, che si sono fatti carico politicamente dell'*iter* del disegno di legge, non sempre facile, nonché ad ISPRA, al suo presidente e all'Associazione delle ARPA, che hanno supportato il lavoro di questi mesi, oltre alle associazioni ambientaliste, a partire dal ruolo svolto da Legambiente. Voglio sottolineare che oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al progetto di riforma ambientale che questo Parlamento sta conducendo come mai prima ha fatto. All'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente e alle norme sulla *green economy* nel collegato ambiente si sommerà positivamente la riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, con la creazione del Sistema nazionale. Altri disegni di legge sono in discussione ed ormai in dirittura d'arrivo, come la riforma delle aree protette, lo spreco alimentare, la Protezione civile, l'acqua, il consumo di suolo. In un clima di crescente preoccupazione riguardo ai temi dell'ambiente, della salute, dei cambiamenti climatici, che la COP21 di Parigi ha riportato al centro del dibattito politico internazionale, è richiesta una risposta da parte delle istituzioni fondata sulla conoscenza, sulla trasparenza, sulla professionalità e sull'etica degli organi tecnici. Solo cosi sarà possibile ridare pienamente quell'autorevolezza indispensabile a riconquistare la fiducia dei cittadini e delle imprese, per farli sentire tutelati nel bene più importante, che è la loro salute, ma anche nell'esercizio della liberta di impresa. Dal 1994, anno della loro costituzione, le Agenzie hanno rappresentato un punto di riferimento per imprese e cittadini, anche se con una risposta non omogenea su tutto il territorio nazionale. Se pensiamo in particolare al Sud del Paese e ai nomi dei siti oggetto di inquinamento e danno ambientale, vediamo manifestarsi concretamente questo squilibrio e questa disomogeneità di trattamento. Questa è un'ingiustizia a cui il disegno di legge in esame pone rimedio, rispondendo concretamente al cosiddetto popolo inquinato del nostro Paese. Il disegno di legge in esame definisce infatti un unico sistema nazionale, superando squilibri regionali e sovrapposizioni normative, indicando nell'ISPRA il polo nazionale e nelle ARPA i poli regionali e territoriali in grado di lavorare in rete, in modo più efficace e omogeneo, attraverso l'attuazione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali Questo sistema dovrà essere l'unico luogo nel quale far convergere e condividere competenze, esperienze, dati e informazioni, attraverso i quali i soggetti pubblici e privati possono trovare un supporto per qualificare, sotto il profilo ambientale, un nuovo sistema di finanziamento sono i principi ispiratori che caratterizzano e qualificano la nuova legge. I cittadini e le imprese dovranno quindi poter contare su un sistema certificato e "terzo" rispetto alle istituzioni, di produzione di dati e analisi sulle matrici ambientali e di relativa informazione ambientale e sanitaria, come già avviene in molte parti del nostro Paese, dopo che è stata svolta anche un'azione di riduzione e di riqualificazione della spesa in tal senso, che non ha sacrificato esperienze e competenze. Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA, definiamo in maniera chiara il rapporto tra controllore e controllato, chiediamo più coordinamento e lavoro in rete, più professionalità a chi dovrà dirigere quelle organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie tra gli enti, che furono anticipate con la con la nascita dell'Associazione delle ARPA nel 2001, come ulteriore tassello verso la costituzione formale del Sistema nazionale. Già il decreto del aveva istituito il Consiglio federale delle Agenzie ambientali quale sede di coordinamento, ma senza sancire, né regolare esplicitamente, l'esistenza e il funzionamento di tale Sistema Solo successivamente, nel 2008, con la nascita di ISPRA questa volontà viene ulteriormente confermata, riprendendo un'organica programmazione delle attività, che dopo una positiva esperienza iniziale, in particolare con i progetti dei Centri tematici nazionali, erano proseguite stancamente e in assenza di una chiara azione di indirizzo. Ora questa esperienza diventa rete vera: dovranno essere messi in rete i numerosi laboratori provinciali e integrate le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determineranno così dei livelli di tutela ambientale di base uguali da Nord a Sud del Paese. Come ci hanno detto i magistrati, impegnati sul fronte delle ecomafie, questo nuovo sistema servirà a rendere più efficaci anche le azioni di repressione entrate in vigore con la legge sugli ecoreati. Concludendo, signor Presidente, ribadisco che anche l'ISPRA in questo disegno assume un ruolo più importante: le 1.306 unità di personale attualmente operanti, attualmente operanti, impiegate ora per l'attuazione del piano triennale, l'espletamento dei servizi ordinari, nonché per le altre attività in convenzione, saranno a disposizione di un sistema nazionale che coordinerà così anche l'attività di ricerca. Questa visione si ricollega al lavoro che il Partito Democratico e il Governo stanno svolgendo anche sul tema del dissesto idrogeologico, del consumo di suolo, della necessità di fornire basi scientifiche per una attenta pianificazione territoriale e, più in generale, nella lotta ai cambiamenti climatici, per meglio applicare la strategia nazionale di adattamento. Oggi, dopo circa otto anni, costruiamo in questo Paese un sistema per la protezione ambientale più forte, dando una organizzazione moderna e innovativa in grado di affrontare le complesse sfide che i tempi attuali ci impongono. Certo, il tema delle risorse non è una questione secondaria, ma grazie anche al nostro ordine del giorno siamo certi che il Ministero e il Governo tutto sapranno corrispondere correttamente e in modo congruo a questa esigenza. Mi auguro tuttavia che, al di là dei pregiudizi verso questo Governo, dei "benaltrismi" sempre presenti, nonché degli eccessi teatrali di alcuni colleghi che abbiamo ascoltato in quest'Assemblea, le forze politiche di opposizione sappiano cogliere qui come alla Camera la specificità e la portata innovativa di questo disegno di legge, condividendo con noi la scelta di approvarlo, inserendo così un altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno e giusto, metta l'ambiente al centro delle politiche di sviluppo per una crescita sostenibile, durevole e inclusiva. È una sfida per tutti che noi vogliamo vincere e non di certo rimandare. Per questi motivi, signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

per esprimere un brevissimo ma dovuto ringraziamento. Nelle varie fasi della discussione è emerso in modo significativo il fattore tempo. Sono stati richiamati più volte i due anni trascorsi dall'approvazione alla Camera ad oggi. Voglio dire che, tuttavia, il provvedimento non è mai stato dimenticato. In questo lasso di tempo, oltre al necessario confronto con il Governo, si è tenuto un vivace e produttivo dibattito con il Ministero, con ISPRA, con AssoArpa e con le associazioni ambientali interessate. A tutti loro va un sincero ringraziamento, così come ringrazio la sottosegretaria Degani e il ministro Galletti per il sostegno politico in questo percorso, tutti i commissari della 13a Commissione ambiente, il presidente Marinello i senatori Caleo e Vaccari che, come Capigruppo del PD, si sono avvicendati in questo periodo, per la tenacia con cui hanno difeso questa riforma, e al consigliere De Salvo per l'assistenza tecnica.

Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla Commissione 12a dopo un approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa. Nel corso dell'*iter* in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (del Governo), 154 (dei senatori Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (dei senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri), 725 (del senatore D'Ambrosio Lettieri e altri), 818 (della senatrice Silvestro e altri), 829 (del senatore Bianco e altri) e 833

è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa. Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di "corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute" (così la relazione d'accompagnamento). Va subito chiarito che la Commissione 12a, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: la proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato durante l'esame in sede referente. Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione. L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali, regolatori ed economici più attrattivi.

prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea sull'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni. I medesimi principi e i criteri direttivi prevedono: l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche; l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, sia su volontari sani, da condurre - e qui c'è la prima novità - con un approccio metodologico di medicina di genere (è la prima volta che nel diritto italiano si parla di medicina di genere); l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse; la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alla domanda per il parere del comitato etico; la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo Inoltre, gli stessi principi e criteri prevedono: la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica; l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche; l'individuazione, nell'ambito degli ordinamenti didattici, di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci; l'aggiornamento periodico; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio; revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali. In sede referente è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la farmacologia di genere. L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di aggiornamento dei LEA e che, sul piano sostanziale, hanno chiarito che il controllo del dolore non deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre, è stato inserito nell'articolo un comma che stabilisce che nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233. Vorrei fare notare che dal 1946 in termini di ordini professionali in campo sanitario non vi è stato alcun aggiornamento. Quindi, questo articolo mi pare di particolare

altri ordinamenti professionali, richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi emendamenti

delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della prevenzione e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente - l'albo della professione di osteopata. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a quest'ultimo ed all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5). In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione - in qualunque forma giuridica svolto, come specificato sede referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo, per la quale sono richiesti il possesso del prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia. Questo significa - lo dico ai colleghi colleghi - andare nella direzione di contrastare in modo sempre più definitivo l'abusivismo professionale. Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale e si sono aggiunte ipotesi di accorpamento. L'articolo 4, L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione dell'osteopata nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti, demandando l'individuazione dei criteri per il

Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia, si prevede che esso sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Spero che questo basti. L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo n. L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. L'articolo 7 modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti. L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in condotte

possano essere definite ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica. In sede referente, è stata operata una correzione di natura esclusivamente tecnica. La novella stati istituiti dalle Regioni). La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un registro *ad hoc* presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel registro,

il comma 1 richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove professioni sanitarie da istituire. L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo. L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province autonome.

Signor Presidente, sinceramente io rimango basita, perché questo è un provvedimento che la Commissione ha

questo provvedimento è in Senato da molto tempo. È stato esaminato attentamente in tutta la fase emendativa dalla Commissione. È iscritto all'ordine del giorno ormai da due settimane e stiamo cominciando a svolgerlo adesso in una forma estremamente ordinata.

sanitari. Se questo non è un ostruzionismo veramente insensato, io non so come altro definirlo. Pertanto, a nome del mio Gruppo, chiedo assolutamente di proseguire l'esame di tale provvedimento. *(Applausi

per ragioni che non sto assolutamente a discutere - raramente è presente, ma sono due anni che stiamo lavorando su questo provvedimento, con la partecipazione di molte persone che, pur non facendo parte della nostra Commissione, ci hanno dato il loro apporto,

con una quantità enorme di audizioni che abbiamo svolto, formali e informali, e che quindi non ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti.

il rischio di quelle malattie che ormai abbiamo dimenticato, che consideravamo debellate, ma che, se si continua ad abbassare questa soglia, debellate non saranno, così come è accaduto in altri Paesi occidentali. l'invito del Ministero della salute, di tanti noi, della Commissione sanità, dei medici pediatri e dell'Istituto superiore di sanità, è quello di dare informazioni corrette. Non è possibile che il servizio pubblico dia informazioni non corrette*.

È necessario che i medici di famiglia, quelli di medicina generale, i pediatri e, ancora di più, noi tutti, insieme, facciamo questo sforzo per spiegare che grazie ai vaccini non si muore più di poliomelite, di difterite e di tetano e di altre malattie e che il vaiolo è scomparso. Questo non è un dato acquisito per sempre: non è che non succederà mai più. Se noi abbassiamo la soglia vaccinale questo spettro potrà ripresentarsi. Che dire poi delle vaccinazioni facoltative? Signori, cari colleghi, la rosolia è una di quelle malattie che, se contratta nella prima fase della gravidanza, determina danni serissimi e gravissimi per la persona, con *deficit* e disabilità drammatiche. Davvero vogliamo scordarci che questo è un problema serio? Davvero dobbiamo pensare che il morbillo è una malattia da bambini? No, il morbillo è una malattia seria, che può complicarsi con problemi gravissimi come l'encefalite. Pertanto, anche se ci possono essere casi rarissimi, eccezionali, collegati talvolta alle vaccinazioni,

Signor Presidente, anche noi vogliamo unirci alle voci che oggi abbiamo ascoltato in Aula di solidarietà nei confronti del Presidente del Parco dei Nebrodi, che è stato vittima di un attentato proprio questa notte. Una Una vera e propria azione di *commando* mafioso, che ha bloccato l'auto su cui viaggiava il presidente Antoci con grossi massi e poi ha sparato all'impazzata contro la vettura. Quest'ultima fortunatamente blindata, lasciato i passeggeri illesi, grazie alla pronta ed efficace reazione degli uomini della scorta che senza esitazione hanno risposto al fuoco, mettendo in fuga i banditi, qualcuno dei quali probabilmente è rimasto ferito perché tracce di sangue sono state riscontrate sul selciato. Si è trattato di un'azione militare che ha visto prevalere gli uomini della polizia grazie al loro coraggio e alla loro dimostrata

Un territorio apparentemente tranquillo, almeno negli ultimi anni, ma che ancora presenta retaggi e rigurgiti dell'arcaica mafia dei pascoli, tradizionalmente organizzata nei territori montani e coraggiosamente contrastata

e imporre la legalità all'interno di un parco protetto; in secondo luogo, di potenziare la vigilanza e la presenza dello Stato in quei territori marginali, montani, difficili da controllare, che richiedono maggiore contrasto alla criminalità, che sembra ben organizzata. Chiediamo al ministro Alfano e a tutto il Governo di fare uno sforzo ulteriore per inviare più uomini e mezzi in quel territorio e per far sì che si possa ripristinare la legalità e la civile convivenza in un'area difficile. Al presidente Antoci, al dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Sant'Agata Militello, dottor Manganaro, che, sopraggiunto sui luoghi, ha partecipato allo scontro a fuoco, in una giornata così difficile va la solidarietà e la vicinanza anche dell'Assemblea del Senato ed un invito a continuare

Signor Presidente, io faccio qualcosa di più che sollecitare delle interrogazioni più e più volte sollecitate. Io richiamo la mozione Amidei e altri, approvata ormai più di un mese fa, con cui il Governo in generale smaltire l'arretrato degli atti ispettivi rimasti senza risposta. Non abbiamo avuto traccia alcuna di alcun cambiamento da parte del Governo, nonostante il voto unanime di quest'Assemblea dato con il parere favorevole del Governo stesso. Allora, se il Governo prende in giro questa istituzione, se il Governo prende in giro questa istituzione, è questa istituzione che deve muoversi e non attraverso burocratici, per quanto sinceri, ma esclusivamente burocratici, inoltri di sollecitazioni. Aggiungo una cosa: visto che ormai da anni una serie di mie interrogazioni sulle questioni delle concessioni autostradali resta totalmente inevasa (non c'è stata neppure una risposta su 11 interrogazioni, ma non è un problema di numeri, avrei potuto presentarne molte di più e mi sono limitato apposta), di più e mi sono limitato apposta), di fronte a tale mancanza di risposte io ho chiesto l'accesso agli atti in base alla legge n. 241 del 1990 e si sono bellamente esauriti i 30 giorni previsti dalla legge stata alcuna risposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Comincio a pensare che ciò che io sospetto, e cioè che ci sia parecchio da nascondere, sia vero. Ora ho presentato ricorso alla Commissione per l'accesso però, francamente, che a interrogazioni parlamentari si debba supplire con la richiesta di accesso, peraltro inevasa e ignorata (non una telefonata e non una riga da parte del Governo) è una cosa inaccettabile e che - e che - ho appreso - avviene esclusivamente nel nostro Paese ed esclusivamente davanti al Parlamento. Tutte le Giunte regionali, provinciali e comunali rispondono a tutte le interrogazioni. I Governi degli altri Paesi rispondono a tutte le interrogazioni. Qui non si risponde neppure ad una richiesta di accesso agli atti.

(le altre sono molte più antiche, ma queste sono aggiornate visto che nel frattempo, grazie al fatto che il Governo non dà nessuna trasparenza, può andare avanti a fare mosse estremamente discutibili) in cui chiedo il contenuto, non l'orientamento o chissà cos'altro, di un protocollo firmato con grande spolvero dal ministro Delrio con amministrazioni locali per cedere per trentun anni una delle più redditizie autostrade d'Italia ad una

qui parliamo di un miliardo e 200 milioni che dovrebbero essere incassati dallo Stato e che invece saranno incassati da una società privata alla quale il Governo ha regalato, regalato, regalato una concessione data in un primo tempo in cambio della realizzazione di una certa infrastruttura che però non verrà realizzata.

finalizzato a far fare un'inaugurazione al presidente Renzi in tempi utili, cioè prima del voto referendario. Questa è una vicenda altresì inaccettabile, perché c'è stata una gara chi l'ha vinta l'ha vinta a determinate condizioni. Visto che l'ha vinta, gli si dà una mancia senza rendere conto al Parlamento (l'abbiamo saputo per caso). La ringrazio, signor Presidente, e chiedo che la Presidenza del Senato si faccia davvero carico di questo, perché non può essere accettabile la semplice trasmissione, una sollecitazione e poi non se ne fa più niente. Sarebbe come se il Senato non mettesse all'ordine del giorno un decreto‑legge del Governo: si deve fare, non è una cortesia. PRESIDENTE. Lo faremo

persone che vivono lì, una piccola comunità caratterizzata da una viabilità che vede un'unica strada che collega il paese, tutt'intorno è caratterizzata da boschi. C'è solo un pulmino che serve per gli studenti. Internet è inesistente e le comunicazioni al cellulare sono molto difficili. Un Paese che di giorno si svuota, perché lavoratori e studenti si spostano; una piccola piazza e un piccolo bar come centro di aggregazione. Ebbene, signor Presidente, in questo contesto si vuole andare ad aprire un centro di prima accoglienza, che dovrebbe ospitare circa una cinquantina di immigrati. I cittadini sono seriamente preoccupati. Si sono rivolti alla prefettura, che ha comunicato la cosa più semplice, cioè che siamo in emergenza e che le persone saranno comunque inviate.

non è certo un posto ideale per avviare processi di integrazione né un luogo dove parcheggiare temporaneamente 48 immigrati. Tengo a precisare, perché la cosa sia estremamente chiara, che i cittadini locali e il gruppo